La seduta è ripresa. Passiamo alla votazione del processo verbale.

nel pomeriggio, in Commissione affari costituzionali dovevamo votare il mandato al relatore sul disegno di legge n. 772, d'iniziativa governativa, sui servizi pubblici locali. Orbene, nel corso della dichiarazione di voto, il senatore Rossi Fernando, riprendendo delle argomentazioni che aveva già sviluppato nel corso della discussione generale, che non avevano trovato accoglimento nel testo uscito dalla Commissione, effettuava dichiarazione di voto contrario. Atteso il numero delle presenze dei senatori della Commissione, era presumibile ed altamente probabile che il mandato al relatore non sarebbe stato conferito. Inutile dire, signor Presidente, che vi è stato un notevole tempo dedicato alle varie dichiarazioni di voto, mentre, attese le presenze e le assenze che si registravano nell'Aula della Commissione, immagino fossero in corso dei conciliaboli. Ciò è assolutamente legittimo, non essendovi dubbio che tra esponenti politici vi può essere un colloquio teso alla convinzione e agli inevitabili ripensamenti. Fino a questo punto, signor Presidente, nulla di strano. strano. Invece, appare davvero stravagante quanto è accaduto poco prima e nel corso della stessa votazione.

il quale non si è limitato ad un intervento di ringraziamento, ma ha ritenuto di utilizzare quel momento per dare delle garanzie al senatore Rossi, nel senso

che per circa un minuto vi fossero 13 mani alzate e 26 occhi rivolti al senatore Rossi, in attesa che quest'ultimo potesse, sia pur timidamente, alzare la mano per conferire il suo voto positivo.

al di là di qualsiasi discorso sui grandi concetti democratici, vorrei dire che effettivamente in tal modo si conferisce al singolo voto una grande pesantezza in ordine

ha ammesso lo stesso senatore Rossi nel corso dei lavori della Commissione, avendo egli affermato che senza quell'intervento non avrebbe votato a favore del provvedimento. Mi lasci anche parlare della particolare lunghezza delle votazioni durante

vera questione è che il problema della democrazia si ancora al rispetto dei Regolamenti, che servono a dare ordine ai lavori delle varie sedute, ma principalmente rappresentano il presidio di garanzia delle opposizioni.

e quindi a spostare l'asse del disegno di legge da una scelta riformista ad una antiriformista.

abbiamo già constatato e constateremo che accadrà - dovesse sposare ancora di più la linea centralista e statalista che la sinistra ha da sempre voluto affermare e che in quest'occasione ha testimoniato con il voto

Debbo dare atto, ringraziandoli per la correttezza assoluta, del comportamento del relatore e del Presidente della Commissione. Il relatore ha preso la parola per 30 secondi - lo voglio dire chiaramente all'Assemblea - per ringraziare

particolarmente importante per il dibattito e il relatore, senatore Sinisi, lo ha voluto sottolineare. Per quanto riguarda poi la

tutti i diritti di cui disponeva; l'ha fatto in un modo chiaro, secondo la prassi della Commissione, alzando la mano. Credo che questo incidente sia artificiale e pregherei i colleghi dell'opposizione di tener conto dell'andamento quotidiano dei lavori di Commissione e, come facciamo tutti da anni, di riconoscere che è giusto che la maggioranza esprima la propria volontà secondo la prassi,

dichiarazioni di voto. Come lei sa, Presidente, e come sanno tutti i colleghi, anche in Aula, io posso parlare quanto voglio; ho la libertà assoluta di votare a favore o contro

parere votando a favore. Si tratta di un qualcosa di politicamente interessante, importante e anche intrigante, se mi consentite. Vorrei sapere che cosa è successo

Sul testo approvato in Commissione, invece, quelle convergenze non si sono trovate perché indubbiamente c'è stato un cedimento, un tornare indietro del Governo accettando le proposte di una parte politica della sinistra estrema che ha sconvolto completamente il provvedimento. Presidente, penso che sia un fatto di costume e di regole; giustamente è stato detto che possiamo bisticciare tra di noi e avere pareri contrari, però, sempre nella correttezza;

ma se diamo anche la sensazione che non siamo seri quando si dice di votare in un modo e poi si vota in un altro, allora, Presidente, ho il timore che le

domenica abbiano messo un po' di tigre nel motore e che, quindi, la spinta propulsiva non si è esaurita e abbiano voglia di sgommare; tuttavia, sarebbe bene che quelle energie fossero dedicate ad altro. Per esempio, potrebbero concordare con le questioni che ho posto in Commissione e cioè che nel progetto Lanzillotta sarebbe bene tener presente il rischio di aumenti dei costi e garanzie per quanto riguarda la qualità dei servizi,

avendo votato anche emendamenti dell'opposizione, come hanno fatto altri componenti della maggioranza in Commissione, così come ho sostenuto emendamenti di Rifondazione e di altri che cercavano di migliorare il testo, che si sia lavorato bene in Commissione. Non guasterei, dunque, un lavoro lungo

intervengo solo per annunciare che fornirò alla Presidenza del Senato - come è giusto e doveroso non solo nei suoi confronti, ma anche nei confronti dei colleghi che hanno sollevato questioni così delicate - ogni opportuno elemento di valutazione, in modo che in una prossima seduta lei possa riferire sulle questioni sollevate. In questa sede, Presidente, vorrei soltanto aggiungere che aggiungere che effettivamente in Commissione affari costituzionali, che svolge un ruolo del tutto peculiare nel Parlamento, al di là della contrapposizione politica tra maggioranza e opposizione, si è lavorato con particolare spirito di attenzione nei confronti delle delicate questioni che sono oggetto d'esame della Commissione.

provvedimenti all'esame della Commissione il rapporto è assolutamente paritario, tanto che la Commissione ha frequentemente relatori che appartengono anche all'opposizione. Mi adopererò in questo senso. Mi consenta una sola osservazione letteraria, visto che il collega Rossi ha citato

Comunque, il senatore Palma ha posto con grande correttezza il problema nel suo primo intervento. Lei, mi ha anticipato, presidente Bianco. Io sono pienamente convinto di due cose: il primo criterio per garantire l'osservanza delle regole della democrazia è il rispetto formale delle regole sempre

sintesi delle diverse sensibilità esistenti sul tema dell'immigrazione, su un aspetto particolare che si riferisce a questo grande tema che ritengo estremamente importante nella società occidentale in genere, che è diventata meta di immigrazione, e italiana in particolare: mi riferisco all'aspetto del contrasto allo sfruttamento dei lavoratori immigrati.

Su questo punto, vale a dire sul contrasto allo sfruttamento dei lavoratori immigrati, e naturalmente allo sfruttamento dei lavoratori in generale, siamo tutti schierati allo stesso modo, cioè siamo fortemente contrari e

Esso, da una parte, contempla sanzioni nei confronti del datore di lavoro e, dall'altra parte, prevede l'estensione anche ai lavoratori colpiti da questa nuova fattispecie di reato di alcune particolari facilitazioni per l'inserimento nella nostra società. Sottolineo

vi è stata la disponibilità da parte dei proponenti e della maggioranza di discutere un testo andando a verificare, parola per parola, provvedimento per provvedimento, comma dopo comma, quali potessero essere le modifiche da apportare alle norme vigenti. un procedimento che ha consentito un lavoro efficace e approfondito, che non lascerà dubbi a chi deciderà di votare il provvedimento perché sa cosa vota. È lo stesso tipo di procedimento che abbiamo usato nella scorsa legislatura per modificare, in generale, le norme sull'immigrazione, con il disegno di legge divenuto la cosiddetta legge Bossi-Fini,

votate molte centinaia di emendamenti per giungere alla fine dell'esame del provvedimento. In quel caso non c'è stata la possibilità di raggiungere un accordo tra maggioranza e opposizione, ma c'è stata la possibilità di vedere con trasparenza e con piena conoscenza di tutti i parlamentari che cosa si andava a votare.

che, invece, risponde a logiche completamente diverse. Tanto per cominciare, è un provvedimento composto unicamente da deleghe - ne ho contate 49, ma, in realtà, siccome alcune sono molto complesse, credo siano ancora di più

secondario rispetto alla logica da cui muove il disegno di legge Amato-Ferrero, che - a mio parere - contrasta anche con la logica del disegno di legge che andiamo ad approvare. Il disegno di legge di cui stiamo parlando è mirato alla

viene punito con pene severe e aggravate nel caso in cui lo sfruttamento sia fatto ai danni di minori di anni 18 o di stranieri irregolarmente soggiornanti, cioè di soggetti che si trovano in situazione di debolezza: i minori di anni 18, di qualunque origine siano,

e di essere privi di sostentamento, con la conseguente possibilità di manifestare disponibilità verso condizioni di lavoro fortemente degradanti, con tutti gli aspetti definiti da questo disegno di legge. un elemento deve essere svolto dal punto di vista della repressione, cioè l'aumento delle pene e anche delle sanzioni accessorie, come per esempio l'esclusione dal percepimento di aiuti dallo Stato o la partecipazione a

sfruttamento. Il disegno di legge approvato nella scorsa legislatura e promosso dal Governo Berlusconi, la cosiddetta legge Bossi-Fini, ha legato la possibilità di entrare e di continuare a risiedere in Italia ad ad un effettivo rapporto di lavoro proprio per evitare che in Italia vi sia un gran numero di persone che si trovino in situazioni di debolezza e di conseguenza portate, per un verso,

di stabilire flussi basati non sulle necessità del mercato del lavoro, ma sulla capacità di assorbimento del mercato del lavoro: se ci sono

di permessi d'ingresso nel nostro Paese perché forse gli altri - quelli che ancora non sono oggetto di richiesta da parte dei datori di lavoro - saranno assorbiti in seguito.

chi avrà un contratto di lavoro da 6 a 12 mesi - cioè anche di 6 mesi e un giorno - potrà restare nel nostro Paese per due anni. E nei rimanenti

che si vuole punire più severamente con questo disegno di legge; dall'altro, essere tentato di infoltire le file della criminalità, una prospettiva di cui i cittadini italiani non sentono davvero il bisogno. Addirittura nel disegno di legge Amato-Ferrero

ma bisogna anche evitare di fornire il serbatoio dal quale trarre nuovi lavoratori da sfruttare e nuove nuove reclute per la criminalità. Mi limito a ricordare una cifra. È noto che un terzo dei detenuti nelle nostre carceri è costituito da persone immigrate nel nostro Paese.

coloro che hanno commesso delitti e sono finiti in carcere sono quasi esclusivamente immigrati clandestini, dal momento che tra gli immigrati regolari il tasso di criminalità è addirittura inferiore a quello medio dei cittadini italiani.

Poiché è altresì noto che gli immigrati clandestini sono particolarmente soggetti a commettere delitti, manifestando un tasso di criminalità superiore agli altri non perché intrinsecamente

pensare di aumentare il serbatoio da cui trarre nuove reclute per la criminalità e tanto meno nuove vittime costrette a lavorare in condizioni inumane e degradanti e dunque gravemente sfruttate. Pertanto, per le stesse ragioni per le quali sono fortemente contrario all'impostazione del disegno di legge Amato-Ferrero, sono favorevole a questo disegno di legge. Su un punto infatti siamo d'accordo: bisogna punire gravemente

È iscritto a parlare il senatore Zuccherini. Ne ha facoltà. Presidente, senatrici, senatori, conoscete tutti la celebre interpretazione di Marx secondo cui la schiavitù funzionò da volano per assicurare un'accumulazione primitiva al nascente capitalismo. La schiavitù era uno dei processi di accumulazione che hanno segnato la nascita dell'era capitalistica. Non siamo in presenza di un ritorno a quella schiavitù storica. La schiavitù, o lavoro forzato contemporaneo, nasce da altre esigenze. Ha origine nei Paesi poveri, in Paesi che hanno visto un crollo repentino delle condizioni di vita. Nasce da guerre esplose in alcune aree; da condizioni di miseria estrema in alcuni Paesi; dall'oppressione delle minoranze; dal disfacimento economico che ha distrutto le precedenti protezioni sociali, seppur minime ed elementari; da crisi che hanno generato spaventose disoccupazioni, definendo un'inedita situazione, perché ha messo in movimento moltitudini di uomini e di donne che premono per arrivare nei Paesi dell'opulenza con il sogno di costruire una vita migliore rispetto a quella drammatica che si lasciano alle spalle. La spinta a migrare sorge anche dal particolare sviluppo economico dei Paesi ricchi, dove la trasformazione della composizione della forza lavoro ha determinato la richiesta di lavoratori a bassa scolarizzazione, provenienti da Paesi poveri e devastati, per lavorare in settori in cui la fatica è una componente centrale del tempo di lavoro. Ci sono aree, zone e spazi economici nei quali il mercato criminale della tratta degli uomini, della riduzione in schiavitù

Secondo uno studio americano commissionato dalla CIA, quindi di una qualche rilevanza, gli immigrati trafficanti in direzione degli Stati Uniti, cioè quelli ridotti in schiavitù o al lavoro forzato, sono almeno 50.000 ogni anno.

L'aspetto più inquietante è che nel XXI secolo milioni di persone sono ancora considerate un oggetto del quale si possa disporre totalmente, perché vengono private della loro autonomia di pensiero, di azione, di movimento. Anche nella civilissima Europa la schiavitù, abolita per legge alla fine del XVII secolo, è oggi una piaga presente più di quanto si possa immaginare. Risulta che i cinesi, che anche nel nostro Paese sono trovati in condizioni di schiavitù e lavoro forzato, in particolare nei settori del tessile e della pelletteria, impiegare anche due anni per raggiungere l'Europa, pagando una somma tra i 5.000 e i 10.000 euro. Alcuni immigrati curdi hanno pagato somme di 6.000 euro per arrivare in Germania. Dalla Repubblica dominicana giungere in Europa costa dai 3.000 ai 6.000 euro. Il traffico di esseri umani rappresenta la più drammatica odierna forma di negazione dei diritti umani

Le persone vengono così trasformate in merce da immettere sul mercato come tante altri merci. Qui sta una delle peculiarità della moderna riduzione in schiavitù. La tratta degli esseri umani appare anche funzionale a un particolare modello del sistema economico. Un recente studio del Fondo monetario internazionale ha evidenziato come il 27 per cento del PIL italiano, prodotto nel triennio 1999‑2001, sia frutto di attività esercitata nel variegato mondo dell'economia sommersa, nel quale sono compresi migliaia di immigrati clandestini, che svolgono lavori spesso rifiutati da tanti nostri connazionali. Tali immigrati vivono in una condizione di lavoro forzato, in quanto sono costretti ad estenuanti orari di lavoro; vengono sottopagati o non pagati affatto; sono privi di coperture assicurative contributive ed obbligati a lavorare e a vivere negli stessi luoghi, in condizioni igienico-sanitarie particolarmente precarie. Simili situazioni sono riscontrabili anche in molti Paesi del mondo sviluppato, lasciando intendere come i nuovi schiavi siano funzionali a un sistema di capitalismo maturo come quello italiano, fondato su una logica neoliberista. La cultura dominante espressa oggi dai ceti oggi prevalenti all'interno del capitalismo italiano e non solo, ritiene che il fine ultimo dell'impresa, ossia il profitto debba essere sempre più basato non tanto sul miglioramento e l'innovazione di processo e di prodotto, ma sulla massima riduzione dei costi della manodopera, dei tempi di produzione e della tassazione. Su un piano più generale, la nuova schiavitù e il lavoro forzato significano dunque grandi profitti per pochi e assenza completa di diritti per milioni di uomini e donne, totalmente esclusi da questa redistribuzione.

del lavoro e del lavoro forzato. Non c'è dubbio che nella formulazione del Governo alcuni passi erano meglio precisati, più espliciti e rendevano più leggibile quella stessa condizione. Nonostante ciò, penso che sia stata raggiunta una mediazione alta

Non c'entra niente la cosiddetta legge Amato-Ferrero, su cui ognuno può avere le proprie opinioni. Noi parliamo della ricostruzione di un diritto fondamentale, della libertà delle persone. Diceva Thomas Paine: «Questi sono i tempi che mettono alla prova le anime degli uomini». Penso che con questa legge si compirà un passo avanti per affermare nuovamente nel nostro Paese un'idea forte della civiltà del lavoro e della condizione

onorevoli colleghi, il disegno di legge, il cui testo ci apprestiamo a discutere, intende promuovere l'adozione di nuove e più efficaci misure di contrasto al fenomeno dello sfruttamento della manodopera di stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale. Con questo disegno di legge, si vuole colpire con durezza il cosiddetto caporalato e l'indegno fenomeno dello sfruttamento lavorativo degli stranieri, che - non può certo sfuggire - in alcuni settori tende a configurarsi come una vera e propria forma di nuova schiavitù. La possibilità, già prevista dall'ordinamento, che allo straniero venga concesso uno speciale permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, quando emergono concreti pericoli per la sua incolumità, viene integrata quindi con una puntuale individuazione della fattispecie di reato per grave sfruttamento di manodopera, i cui requisiti ricordo brevemente: retribuzione retribuzione ridotta di oltre un terzo rispetto ai minimi contrattuali; sistematica e grave violazione della disciplina in materia di orario di lavoro e riposo settimanale; gravi violazioni dei requisiti di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, con esposizione dei lavoratori a elevati rischi per la loro salute, sicurezza e incolumità; reclutamento e avviamento al lavoro secondo le modalità che vengono comunemente indicate con il termine di caporalato. L'iniziativa ha lo scopo specifico di aggredire una grave patologia del sistema produttivo, lo sfruttamento della forza lavoro che, attraverso attività lesive dei diritti fondamentali della persona, crea economie illegali, ostacola la concorrenza e falsa gli equilibri di mercato. L'alto livello di irregolarità dei lavoratori extracomunitari nel territorio nazionale è del tutto connesso alla forte incidenza dell'economia sommersa: sommersa: sanzionare la prima significa incidere sulla seconda. Non può essere dimenticato che l'intermediazione e la somministrazione abusive di manodopera si traducono fin troppo spesso in forme di sfruttamento e violenza, che configurano talvolta una vera e propria riduzione in schiavitù, di cui sono vittime soprattutto lavoratrici e lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno. Sotto questo

della manodopera extracomunitaria, particolarmente vulnerabile quando versa in condizioni di irregolarità. Tuttavia, un esame attento del disegno di legge nel suo complesso non può non sollevare perplessità sul modo in cui si intende perseguire questo fine. di sfruttamento, secondo il presente testo, davanti ad una retribuzione ridotta di oltre un terzo rispetto ai minimi contrattuali previsti dai contratti collettivi di categoria, a gravi violazioni della disciplina in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e a forme di reclutamento e avviamento al lavoro secondo modalità irregolari.

a immigrati clandestini, ovvero allungando i tempi per i regolari (il permesso per i lavoratori stagionali dura nove mesi, mentre quello per motivi di protezione sociale dura diciotto La nostra preoccupazione è che, sfruttando questa norma, ci possa essere un giro di prestanome per arrivare alla regolarizzazione dei clandestini. Gli effetti del disegno di legge potrebbero essere drammaticamente controproducenti, perché si potrebbe indurre l'immigrato irregolare a simulare condizioni di sfruttamento allo scopo di strappare un permesso di soggiorno, oppure si potrebbero creare imprese di comodo, ditte virtuali, per non dire fasulle, magari intestate a prestanome anziani e nullatenenti, allo scopo di assumere in modo fittizio dipendenti da fare poi emergere, ponendo il titolare in qualche modo al riparo da eventuali sanzioni. Ai colleghi senatori non può sfuggire che la materia dell'immigrazione, inoltre, va trattata con equilibrio e discernimento, tenendo presenti tutte le disposizioni legislative in vigore. La repressione dello sfruttamento del lavoratore irregolare non può prescindere da tutto il contesto non solo normativo, ma anche sociale ed economico, che ha portato una persona extracomunitaria a trovarsi irregolarmente sul nostro territorio, dove è costretta poi ad accettare condizioni di lavoro incompatibili con la dignità umana. Sebbene sia lodevole l'intenzione che muove questo disegno di legge, le prescrizioni in esso contenute sembrano muoversi in una direzione confliggente con il panorama normativo oggi in vigore, se non in termini espliciti, sicuramente dal punto di vista di una aggirabilità dei suoi effetti. E questo, come fin troppo spesso ormai accade, attraverso l'emanazione di norme che, sebbene mirate e puntuali nella singola fattispecie, rischiano di scardinare l'intero orizzonte normativo in cui dovrebbero invece inserirsi. Mi chiedo, infatti, come sia possibile coniugare lo spirito di questa legge con quello delle norme contenute nella legge Amato-Ferrero sull'immigrazione, che aprendo le maglie all'ingresso favoriscono la permanenza sul nostro territorio in assenza di lavoro, e quindi rischiano di incentivare l'attività di caporalato; anche perché - giova precisare, e questa forse sembra la peggiore mancanza del testo - questo disegno di legge affronta la materia solo dal lato della repressione, ma dimentica l'altro, quello dello sviluppo di una cultura della prevenzione. In questa sede non può essere dimenticato, infatti, come esistano nella pratica quotidiana evidenti fenomeni di vera e propria complicità tra gli sfruttati e gli sfruttatori. Senza una puntuale analisi delle logiche sottese, non è evidentemente possibile sostenere di aver inquadrato, compreso e affrontato completamente il fenomeno. La confusione e la fretta spesso portano a tradire le aspettative a tutto discapito delle buone intenzioni; un errore che non ci possiamo permettere, soprattutto in un momento in cui la classe politica non gode certo di un eccesso di fiducia. Oggi l'eccessiva presenza di immigrati sul territorio è fonte di insicurezza diffusa nei nostri concittadini. Rischiare di provocare un aumento indiscriminato della presenza di extracomunitari, ovvero anche solo darne l'idea, alimentarne il sospetto sembra contribuire ad una polarizzazione sociale della comunità nazionale che il recente voto amministrativo ha già posto in luce; soprattutto, genera una preoccupazione che rischia di offuscare e sminuire le comunque lodevoli intenzioni di questo disegno di legge.

Signor Presidente, capisco che potrò anche commettere un peccato di presunzione, che è a metà tra un peccato veniale e un peccato più grave, anche se non un peccato mortale, e chiederò a qualche collega poi di difendere le mie sorti, perché possa essere pienamente difeso rispetto alla condanna che me ne può derivare come disattenzione o come elaborazione di tesi contrarie alla mia. mia. Io, contrariamente a molti interventi di questa parte politica, non sono assolutamente d'accordo sul provvedimento in esame, non perché non ritenga valida la proposta che viene fatta, ma per quanto ho argomentato in Commissione bilancio, cioè

del Senato, il quale dispone: «Sono assegnati per il parere alla 5a Commissione permanente i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate o che contengano disposizioni rilevanti ai fini delle direttive e delle previsioni del programma di sviluppo economico».

nelle Commissioni di merito 1a e 11a riunite e che l'Aula dovesse valutare, vista la pesantezza, il parere della Commissione bilancio. Perché dico questo? Signor Presidente, non ritengo oggi che noi si sia alle porte di un nuovo 7 ottobre 1571. I colleghi ricorderanno che il 5 ottobre del 1571 è il giorno al quale, pur con i cambiamenti del calendario, si fa riferimento per la battaglia di Lepanto, che fermò, secondo alcuni, un processo di novella migrazione rispetto a quella che (anche se esaminata da tanti libri di storia come una migrazione dei popoli orientali verso l'Occidente) per tanto tempo gli storici e gli studiosi di economia hanno valutato non fosse una vera e propria migrazione, ma una emigrazione. Gli arabi - che si trovavano in Spagna e in Italia - non avevano dato atto ad una migrazione, ma ad una emigrazione, poiché vi si erano stabiliti militarmente e quella che nei testi di storia viene presentata come una collaborazione tra diverse popolazioni di fatto era la presenza di popoli arabi

per l'aumento della popolazione d'Occidente, conseguente alla soluzione dei problemi sanitari in terra d'Occidente, ad una impossibilità di ricevere quella migrazione che si era cominciata a presentare agli albori rinascimentali. Gli albori rinascimentali, facevano sì, con le teste di ponte costituite dalla prime emigrazioni orientali, che la migrazione venisse ad essere attratta dalle nuove condizioni economiche dell'Occidente. Oggi ci ritroviamo nelle stesse identiche situazioni, con con una situazione economica, cioè, di gran lunga "migliorante", nel senso che migliora con una velocità enormemente superiore nelle terre d'Occidente e in alcune aree delle terre orientali, edin questo senso si ha uno spostamento di popoli. Ora, non essendo possibile una nuova battaglia di Lepanto (non

la presunzione di questo Governo, di codesto disattento Esecutivo seduto ai banchi del Governo? Non me ne vorrà l'amico Franco Danieli, che è l'unico rappresentante che potrebbe, per la sua preparazione, prestare un minimo di attenzione

La presunzione della "Bossi-Fini" era quella di cercare di valutare un fermo alla trasformazione dell'emigrazione in migrazione. Questo Governo, dicendo che quel sistema non aveva funzionato, ha detto qualche mese addietro che avrebbe presentato un nuovo disegno di legge, cioè l'Amato-Ferrero. Non il Ferrero in quanto amato; Amato è il Ministro, poi vi è un Ferrero. Il Ferrero da noi non è affatto amato. Amato è amato per i fatti suoi!

riformato con un decreto-legge; pertanto, non potendo procedere con un provvedimento d'urgenza, è stato presentato un disegno di legge. Pertanto, in attesa di un disegno di legge annunziato, di cui non si conosce il contenuto,

necessario. È assolutamente necessario che il provvedimento sia inserito nel contesto della programmazione complessiva, con riferimento alla necessità di salvaguardare il nostro Stato, la nostra Nazione, le nostre Regioni e le nostre attività economiche dalla migrazione, perché un riferimento

è un errore politico madornale presentare sotto campagna elettorale questo provvedimento, spacciandolo come l'attesa riforma della Bossi‑Fini e quindi anticipando il contenuto della Amato-Ferrero

un normale*iter* in Commissione bilancio, tant'è che la Commissione si è trovata in difficoltà nel dover esprimere il parere. Se viene letto con la dovuta attenzione, come sono sicuro che hanno fatto i componenti del Governo oggi presenti in Aula e i colleghi della maggioranza che se ne sono occupati,

riserve sui contenuti propri del provvedimento, che potrebbero essere meglio affrontati - come ha più specificatamente e dottamente argomentato il collega Malan poc'anzi

il Senato sta esaminando in Aula un disegno di legge che è già superato

che pone all'attenzione del Parlamento le norme oggi in discussione (modificate, certo, dal lavoro svolto nelle Commissioni riunite), in epoca successiva di qualche mese

che modifica completamente l'intero testo unico sull'immigrazione, anche nella parte relativa al grave sfruttamento degli immigrati extracomunitari. Questo credo richieda una riflessione, intanto dal punto di vista formale, poi anche da quello sostanziale. La modifica sulla quale il Governo chiede al Parlamento una delega, per poi intervenire con norme di dettaglio, riguarda disposizioni originariamente prese in considerazione dal disegno di legge in discussione (penso all'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione)

non è ancora stato assegnato al Parlamento; non so se lo sia stato nelle more tra la discussione delle Commissioni riunite e l'Aula. Può darsi che non sia stato ancora svolto il passaggio nella Conferenza Stato-Regioni. Tutti noi, però, sappiamo - e, se non lo sappiamo, basta consultare l'aggiornatissimo sito del Ministero dell'interno che questo disegno di legge esiste, non è un annuncio, e che, articolato e messo per iscritto in modo abbastanza puntuale, è stato approvato dal Consiglio dei ministri.

oggi il Parlamento prendere in esame delle norme che incidono su alcuni settori del testo unico sull'immigrazione, posto che lo stesso Governo ha varato al Consiglio dei ministri - e quindi tutti noi abbiamo avuto la possibilità di leggerlo - un articolato che modifica anche quelle disposizioni? Si dirà Si dirà che questo è vero solo in parte, perché correggendo, a seguito del lavoro svolto dalle Commissioni riunite, l'impostazione originaria, il riferimento che all'inizio c'era all'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione oggi diventa una nuova norma del codice penale. Quella nuova norma però contiene, anche dal punto di vista lessicale, elementi di assoluta sovrapposizione con l'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione, e comunque si interseca con quella disciplina

una delega ampia, onnicomprensiva, fondata sull'assunto ideologico, che non riguarda soltanto la materia dell'immigrazione, in base al quale fino al

proporre al Parlamento un'intera riscrittura del testo unico sull'immigrazione, che senso ha questo acconto, questa anticipazione, che si tradurrà inevitabilmente in un doppio lavoro da parte del Parlamento? È vero che il Parlamento non sta lavorando o sta lavorando molto poco, ma non è il caso che si eserciti o che faccia delle anticipazioni su ciò che non costituisce anticipazione ma che ad un'iniziativa legislativa già approvata dal Consiglio dei ministri, tant'è che chiunque, attraverso internet, può coglierne ogni passaggio. Nel merito, queste disposizioni costituiscono uno strano *mix* tra violazioni del diritto penale già coperte da sanzione, violazioni del testo unico sull'immigrazione già coperte da sanzione, violazioni delle disposizioni contrattuali che trovano una via non penalistica di soluzione attraverso il ricorso al giudice del lavoro. Questo *mix* che viene realizzato ha un tasso di genericità, di contraddittorietà e di indeterminatezza che renderà molto difficile all'interprete capire quale sarà la norma cosiddetta speciale da applicare nel caso concreto. Mi limito al primo comma del nuovo articolo 603-*bis* del codice penale introdotto dall'articolo 1 di questo disegno di legge. recita: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque» - vediamo quale è la condotta - «recluti lavoratori, ovvero ne organizzi l'attività lavorativa» viene poi il come - «sottoponendo gli stessi a grave sfruttamento». Quindi, la condotta essenziale si sostanzia in un grave sfruttamento; le modalità di questo grave sfruttamento sono: o la violenza - ci sono delle virgole, quindi delle disgiuntive

da gravi violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale, connesso alla organizzazione e gestione delle prestazioni, gravemente degradante, La norma è scritta - lo ripeto - in modo confuso, con poca punteggiatura, per cui il rischio di interpretazioni poco chiare c'è tutto. In questo rischio si inserisce anche l'ipotesi che una differenza salariale significativa possa costituire indice, anche implicito, anche indiretto, di minaccia o di intimidazione. Mi è capitato più volte, signor Presidente, svolgendo le funzioni di giudice penale, di trovarmi di fronte a contestazioni di estorsione in di trovarmi di fronte a contestazioni di estorsione in presenza di notevoli differenze salariali accompagnate da intimidazioni e da minacce anche implicite. sufficiente non minacciare direttamente il licenziamento, ma farlo in qualche misura comprendere. Ora, noi introduciamo una norma in una parte del codice penale in cui ci sono reati gravissimi odiosi. Non dico che lo sfruttamento dei lavoratori non sia grave e odioso, ma che stiamo introducendo questa norma in una parte del codice penale che contiene sanzioni per la tratta di schiavi che c'è il rischio che si qualifichi come tratta di schiavi una pratica, certamente non gradevole e da sanzionare con gli strumenti previsti dall'ordinamento, ma che in qualche caso può essere esclusivamente una controversia per differenze salariali. Vogliamo mettere la sorte di aziende che vanno sanzionate - e nella legislazione vigente esistono le norme per punirle nelle mani di denunce che in qualche caso possono essere strumentali, ma che in via cautelare possono portare al blocco dell'attività di queste aziende? È un rischio che deriva dalla formulazione - ripeto - poco chiara, confusa di questa norma. inoltre, di condizioni degradate: basterà ogni violazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per attivare questa disposizione penale? So che il Governo o il relatore risponderanno di no, però l'articolazione della norma è tale che, perlomeno come ipotesi iniziale d'indagine, un'iscrizione nel registro degli indagati per questo tipo di reato ci può essere e, in via cautelare, questa ha effetti diretti non soltanto sull'azienda, ma anche sugli altri lavoratori di quest'azienda. Credo che la casistica giudiziaria sia piena di denunce, anche penali, che sorgono quando l'animosità tra il lavoratore e il datore di lavoro è tale che non ci si accontenta del ricorso al giudice del lavoro e la denuncia penale diventa uno strumento per rafforzare, appunto, il ricorso al giudice del lavoro. In realtà, questo disegno di legge sconta un'ambiguità originaria perché inizialmente era stato costruito attorno ad una dilatazione dell'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione,

Quella norma ha una struttura, una finalità e un oggetto specifici, nel senso che riguarda la tratta di esseri umani e la la moderna riduzione in schiavitù che passa attraverso la lacerazione di vite di giovani donne moldave, ucraine, rumene o di altra nazionalità che vengono prelevate nel loro Paese dai

non soltanto l'immediata attivazione dell'indagine penale, ma anche, uno specifico programma di protezione a tutela del denunciante che può diventare anche testimone. Questo programma di protezione non riguarda soltanto strette cautele di sicurezza, ma prevede un inserimento di chi denuncia nel contesto sociale e legale italiano, con un permesso di soggiorno per studio o per lavoro, se l'extracomunitario che viene tirato fuori da questo giro sceglie questa seconda strada, il ritorno assistito nel Paese di origine con una sorta di borsa lavoro o borsa studio che gli consente una reimmissione nel Paese di origine. Ora, chiedo a lei, signor Presidente, al Governo e al relatore Se stiamo parlando di grave sfruttamento e quindi si riprende testualmente la terminologia contenuta nel testo unico sull'immigrazione all'articolo 18 per la tratta di esseri umani

la previsione, per chi denunci un grave sfruttamento ai sensi del nuovo articolo 603-*bis* del codice penale, di un programma di protezione? Forse che chi denuncia una sorta di tratta di lavoratori extracomunitari non rischia come la ragazza diciottenne o sedicenne che denuncia i suoi sfruttatori? Per quale motivo, in queste disposizioni, manca un richiamo anche formale a quella parte dell'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione che tutela concretamente? E quante centinaia di testimoni e di denuncianti sono stati tutelati. Non vorrei che quest'assenza dipendesse da quella carenza di fondi oggi denunciata nell'altro ramo del Parlamento dal ministro Amato, visto che si parla di svariate centinaia di milioni di euro. Ma se manca la possibilità materiale di far fronte alla tutela dei denuncianti di un reato così grave e odioso, forse è il caso di lasciare in piedi la legislazione vigente, che appresta una tutela meno confusa e più specifica con riferimento alle varie ipotesi di reato. Credo che nessuno in questo Parlamento, in questo Senato, abbia neanche la più remota idea di collusione o di complicità con chi sfrutta i lavoratori, italiani o stranieri,

certo ricordarlo a lei. Ci sono gli ispettori del lavoro: verrebbe da chiedersi perché non sono andati a svolgere ispezioni nei campi di raccolta del pomodoro del foggiano o del salernitano che si vedono, transitando sulle autostrade.

Perché rendere più confuso il quadro normativo? Tale quadro normativo che verrebbe reso ancora più precario se questo disegno di legge delega, il cosiddetto Ferrero-Amato, dovesse essere, un giorno, approvato. disegno di legge delega che ipotizza l'abolizione del contratto di soggiorno e che consente l'ingresso nel territorio nazionale anche a chi non ha un contratto di lavoro o un'ipotesi di contratto di lavoro e deve cercarlo: il che significa, nelle more della ricerca e in presenza di un fondo di garanzia che, certo, è previsto nel disegno di legge delega, ma è inimmaginabile che possa essere sufficiente a mantenere tutti gli stranieri che entreranno per ricercare lavoro, diventare facile preda dello sfruttamento in nero, se non, in una parte marginale, della tentazione della criminalità. Vorrei tanto, signor Presidente, che il Senato svolgesse un'attività legislativa più consistente, più serrata di quella che ha esercitato da un anno a questa parte, però ritengo veramente paradossale che, nel momento in cui decide di legiferare, lo faccia su materia sulla quale lo stesso proponente del disegno di legge in discussione, vale a dire il Governo, annuncia in epoca successiva una revisione completa che riguarda anche la materia qui in esame. Sulla base di questo paradosso,

per cui se la definizione generale può essere intesa in un certo modo e per esempio è condivisibile, poi il contesto ideologico in cui è inserita e la finalità non dichiarata sono esattamente l'opposto Per essere chiari, è ovvio che la Lega assolutamente condivide il principio che nessun essere umano deve essere volontariamente sfruttato, né nell'ambiente di lavoro né in qualunque altro ambiente, ed è ovvio che siamo per definizione per l'assoluta legalità dei rapporti di lavoro di qualunque tipo; tant'è che questi, anche nel caso dell'immigrazione, sono esattamente i princìpi contenuti nella legge Bossi-Fini, che lega la gestione razionale del fenomeno migratorio proprio a questi princìpi e a queste questioni, quindi alla possibilità di dare un lavoro regolare e decoroso alle persone che vengono nel nostro Paese, più tutta una serie di altre garanzie per le persone stesse. Ovviamente, siccome i princìpi devono poi essere accompagnati da prassi ragionevolmente utili al perseguimento dei princìpi stessi,

come per esempio la dichiarazione di una persona attendibile che fornisca la casa, un contratto di lavoro per cui la persona viene in Italia non sulla parola ma su un dato di fatto in qualche modo consolidato. Se parliamo di queste cose, è ovvio che siamo assolutamente d'accordo con quanto viene enunciato anche qui come principio. Detto questo, dobbiamo però inevitabilmente fare una serie di distinguo distinguo che sanzionano la differenza di impostazione ideologica che c'è tra noi e i proponenti il provvedimento.

ma è uno dei tanti fenomeni che hanno a che fare con la vita pubblica dei Paesi, in particolare del nostro e dei Paesi occidentali simili al nostro, che per definizione chi amministra la Nazione - quindi i politici, gli eletti dal popolo - deve affrontare in maniera ragionevole, razionale, intelligente, il tutto possibilmente finalizzato al benessere complessivo dei cittadini rappresentati e della popolazione del resto del mondo. Il fatto che sia un fenomeno assolutamente gestibile lo dimostrano i Paesi che lo gestiscono, perché le cose che succedono in Italia non è che succedono in tutti gli altri Paesi del mondo,

non esistono in Francia, che ha una presenza di immigrati più elevata della nostra ma per ragioni storiche precise, anzi per molti anni c'è stato uno scambio assolutamente normale considerato la situazione coloniale in cui viveva quel Paese; non è così in Spagna,

le sanzioni e le modalità di gestione dell'immigrazione sono enormemente diverse dalle nostre. Per non parlare poi, paradossalmente, dei Paesi da cui provengono

inevitabile e incontrollabile. È piuttosto una scelta. Quindi, se è controllabile, dipende poi dalla politica, dall'impostazione strategica che si dà alle scelte politiche,

provvedimento si basava su princìpi estremamente semplici e chiari. Il nostro Paese è disponibile ad accettare un certo numero di persone provenienti da altri Paesi, ma ciò è legato esclusivamente alla possibilità e disponibilità di posti di lavoro, alla necessità degli stessi e comunque il tutto dev'essere fatto in modo da essere compatibile per la società che accoglie - l'Italia - e decoroso per le persone che vengono da noi, vale a dire gli immigrati.

di trovarsi in una situazione di irregolarità, nel senso che, per definizione, le persone che fossero entrate nel nostro Paese rispettando la legge Bossi-Fini avrebbero seguito un percorso di perfetta legalità. Anzi,

normale, razionale, kantiano, in cui ad una causa segue un effetto e un qualcosa in mezzo che fa funzionare le cose. Nella vostra volontà di smantellare qualsiasi cosa sia stata fatta dal centro-destra

prevederebbe l'invasione tranquilla e garantita da parte degli organi istituzionali dello Stato, del nostro Paese da parte di chiunque ci voglia entrare.

quote. Mi piacerebbe capire, da un punto di vista puramente logico, come fate a giustificare l'immigrazione con l'esigenza lavorativa del nostro Paese e poi togliere ogni riferimento alle quote.

senza che seguano una programmazione dello sviluppo economico, qualcuno mi deve spiegare come potete poi legare l'ingresso di queste persone alla necessità lavorativa, come pure sempre fate, quando parlate di queste questioni. Dirò di più, che senso ha fare un provvedimento come questo, che sanziona in maniera precisa, anche giusta per tanti aspetti, quasi feroce in alcuni passaggi, chi non rispetta le regole di rapporto contrattuale tra datore di lavoro e lavoratore, in questo caso l'extracomunitario, quando voi siete i primi ad incentivare questa situazione e questa prassi? È ovvio che se introducete quantità enormi di persone

l'ingresso illegittimo è di per sé un reato, quindi incentivate le persone ad entrare illegalmente, a commettere un reato. E dopo che avete messo sul piatto l'occasione per i cittadini altri

neanche tra l'italiano, bensì tra l'occidentale capitalista sfruttatore (l'abbiamo visto in qualche intervento che richiama ancora le ideologie del secolo scorso che hanno causato 80 milioni di morti per fame e miliardi di persone schiave del lavoro) e

Il grosso del caporalato in edilizia non è più rappresentato dal calabrese o dal siciliano o comunque dall'italiano che va sulla piazza e raccoglie i poveracci del Paese, ma tra loro

Noi in Italia siamo capaci di infliggere milioni di euro di multa a chi sbaglia un codice fiscale su una bolla di accompagnamento regolare e poi abbiamo delle situazioni veramente da Terzo mondo, rispetto alle quali si chiudono gli occhi perché loro sono dei poveracci.

è evidente che noi non ci possiamo assolutamente trovare d'accordo con voi; non possiamo minimamente condividere questo vostro modo di ragionare. ragionare. Ci piacerebbe altresì capire quale sia, alla fine, la posizione vera del Governo, della maggioranza o chiamate come volete il gruppo di persone che in questo momento governa il Paese. È quella di Prodi che va a stringere la mano a Zapatero per concludere un accordo bilaterale sulla difesa dei confini contro l'immigrazione clandestina?

che in Italia debba entrare chiunque lo voglia, perché è giusto così e non è assolutamente giusto bloccare i flussi migratori, perché questo è il destino del mondo.

Queste sono dichiarazioni ufficiali pubblicate sui giornali da parte del ministro Ferrero. Qualche settimana fa, avendo un attimo di tempo, ho ritrovato un libercolo del secolo scorso

dimostrando il suo grande attaccamento al Paese e all'Occidente, ha fatto anche delle altre uscite di un certo rilievo, che lo pongono nell'alveo dei grandi statisti, dichiarando che un italiano da zero a 18 anni costa 150.000 euro quindi è meglio prendere un extracomunitario già adulto, in modo da risparmiare soldi. vostra impostazione mentale è questa, è ovvio che, anche se queste poche righe sono condivisibili perché è il nostro modo di pensare (l'immigrazione si regola con i rapporti di lavoro regolari), è ovvio che tutto il contesto ideologico in cui voi la inserite non è assolutamente condivisibile.

sui tanti aspetti che sono stati sollevati dai colleghi dell'opposizione e della maggioranza. Mi limito innanzitutto a ricordare che sul provvedimento in discussione c'è stata piena convergenza in Commissione. Questo è già un fatto molto importante. Rilevo che molti interventi dei colleghi dell'opposizione sono stati sostanzialmente, e anche formalmente, in favore di questo provvedimento e ciò mi rallegra assai.

storico-politica, economica, sociale sulle origini dell'immigrazione, sulla spaccatura del Mediterraneo dopo la battaglia di Lepanto, sopra le origini della schiavitù, il modello capitalista,

mi limito a registrare appunto la sostanziale convergenza sugli aspetti di questo particolare provvedimento, che riguarda il contrasto alle gravissime situazioni di sfruttamento, molto spesso vicine a forme di schiavitù, fatti i dovuti collegamenti temporali, i dovuti paragoni e i dovuti sconti. su questo provvedimento mi sembra che ci sia un sostanziale accordo. Certo, non raccolgo nemmeno tutte le indicazioni che sono state sul possibile contrasto procedurale tra questo provvedimento e la futura legge delega sull'immigrazione. Credo che il collega Bianco lo farà per me. Quindi ringrazio tutti gli intervenuti. Credo che questo sia un buon provvedimento, che viene al momento opportuno. Nessuno pensa che l'Italia sarà un Paese sommerso dall'immigrazione, ma per fare questo bisogna elaborare buone leggi, bisogna ridurre al massimo il sommerso, che è una delle grandi piaghe del nostro Paese, perché è l'economia sommersa, l'economia in nero che attira l'immigrazione, e certamente nel futuro bisogna ristrutturare anche la nostra economia. Una economia con più tecnologia e meno intensità di lavoro sarà un'economia che richiede meno immigrazione. Certamente questo è vero, ma si tratta di obiettivi di lunghissimo periodo che trascendono il termine della nostra discussione. Ringrazio tutti per l'attenzione. Signor Presidente, rispondo telegraficamente a due osservazioni specifiche che sono state mosse nel corso del dibattito, la prima delle quali dal collega Ferrara riguardo al parere della Commissione bilancio. Le Commissioni riunite e i relatori hanno tenuto conto ovviamente del parere della Commissione bilancio, che è un parere favorevole, non ostativo. Quindi, obiettivamente il dibattito interno attraverso cui si arriva a questo parere non ha alcun rilievo al di fuori della Commissione. Ripeto, il parere della Commissione bilancio è un parere non ostativo. Per quanto riguarda la seconda questione, sollevata in particolare dal collega Mantovano (egli l'aveva già sollevata in Commissione), essa è relativa ad un potenziale conflitto con un altro provvedimento. Sottolineo che il provvedimento in oggetto non è ancora stato presentato in nessun ramo del Parlamento; risulta approvato dal Consiglio dei ministri, ma è all'esame della Conferenze unificata. Comunque, siccome si tratta di un rilievo serio, lo abbiamo esaminato esaminato con grande attenzione nelle Commissioni e abbiamo chiesto al Governo se riteneva che ci fosse una potenziale sovrapposizione tra i due provvedimenti. Il Governo ha affermato che mantiene l'intendimento di proseguire l'esame di questo disegno di legge ed è la ragione per la quale abbiamo ulteriormente lavorato. Vorrei sottolineare, signor Presidente, come ha fatto il relatore Livi Bacci, che anche dopo questi rilievi, le Commissioni hanno lavorato in modo molto proficuo e il provvedimento è stato approvato con la sostanziale unanimità da parte delle Commissioni riunite 1a e 11a, naturalmente nell'ambito del distinguo politico in cui è stato comunque presentato. PRESIDENTE.

anche se non è lo stesso che il Governo ha presentato, ne riprende le ragioni e le finalità; soprattutto è un testo apprezzabile proprio perché è il frutto di un approfondito dialogo che c'è stato nelle Commissioni e che ha consentito, nella redazione, di trovare un punto d'incontro politico che rappresenta anche la forza di un intervento di contrasto allo sfruttamento dei lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale. Vorrei dire anche che, con riferimento alla legge sull'immigrazione, sia che ragionassimo nell'ottica della legislazione attuale, sia che ragionassimo nell'ottica di una possibile riforma, qui vogliamo invece aggredire una grave patologia del sistema, in particolare del sistema produttivo, che è lo sfruttamento della forza lavoro; un fenomeno che, attraverso attività lesive dei diritti fondamentali della persona, crea delle economie illegali, ostacola la concorrenza e falsa gli equilibri del mercato. Ho sentito dire nella discussione che, attraverso questo sistema, sia anche possibile un equilibrio nell'incontro fra domanda e offerta. Credo si tratti di un equilibrio apparente per gli effetti deteriori ed iniqui che produce nel breve e nel medio periodo, nocivo alla convivenza sociale ed allo sviluppo economico; avversario proprio di quelle regole che ciascuna parte politica, indipendentemente dalle proprie impostazioni intende affermare in materia di immigrazione regolare. Voglio solo richiamarvi a leggere la relazione che ha curato il CESIS, dove a proposito del contrasto alla gestione criminale dell'immigrazione clandestina, evidenzia una capacità organizzativa dei traffici, tale da garantire anche lo sfruttamento della manodopera e di intercettare i circuiti finanziari delle rimesse. Si dice che nei circuiti di sfruttamento in quella relazione sovente si produce una vera e propria riduzione in schiavitù, supportata dal sistematico ricorso all'intimidazione ed alla violenza. Un fenomeno ampio, nel quale vengono coinvolti a volte soggetti criminali, a volte piccoli imprenditori estranei alla tratta, ma disponibili a sfruttare i lavoratori, siano essi clandestini o regolari. Vorrei anche tener conto, e lo avete fatto nel testo, che l'intermediazione abusiva, il cosiddetto caporalato, così come la somministrazione abusiva si declinano a volte con modalità di sfruttamento e di violenza, con soprusi che descrivono anche essi forme di riduzione in schiavitù. Ci è evidente anche il dato dalle indagini delle Forze di polizia che i soggetti che subiscono di più sfruttamento del lavoro sono proprio gli immigrati, gli extracomunitari ed in particolare quelli privi di permesso di soggiorno. Per questi la condizione di irregolarità diventa condizione di vulnerabilità, di soggezione, di dipendenza, anche perché gli è impossibile agire quelle tutele che farebbero anche emergere la loro clandestinità con le relative conseguenze. Così come non mancano immigrati che in questo contesto si trasformano da vittime in sfruttatori di altri immigrati. Più l'economia sommersa si alimenta della manodopera straniera, più la sua offerta attrae immigrati e produce immigrazione clandestina, più si realizzano meccanismi perversi di sfruttamento. Credo che questo testo risponda un po' alle esigenze e alla rappresentazione della realtà che insieme agli organi di polizia ci danno gli organi di stampa. Voglio solo aggiungere, interloquendo con l'intervento del senatore Mantovano, proprio in considerazione di osservazioni avanzate sia dalla maggioranza che dall'opposizione con riferimento all'articolo 18 la scelta della Commissione, che il Governo ha condiviso, è stata quella di non toccare l'attuale formulazione di tale articolo, nella quale la previsione penale che stiamo introducendo entra soltanto perché per il carattere della pena e per previsione espressa rientra tra le fattispecie di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale. Vorrei anche dire al senatore Mantovano che sa bene che non è solo la previsione della tratta quella attualmente considerata dall'articolo 18, ma sono proprio quelle forme di sfruttamento che possono ricavarsi anche nelle disposizioni in quei reati stabiliti dallo stesso articolo 380 del codice di procedura penale. Anche questo caso quindi, come quegli altri,

di ottenere un permesso di soggiorno, qualora corra seri pericoli per la propria incolumità nel tentativo di sottrarsi da una organizzazione criminale. Dico anche che il disegno di legge delega che il Governo ha in mente e che il senatore conosce bene ma credo sia abbastanza diffuso intende intervenire non sui soggetti

pur non correndo un pericolo lei stessa, si trovi ricattata o minacciata per l'incolumità dei suoi familiari che magari sono rimasti nel Paese d'origine. Credo che questi temi, davvero come hanno vissuto nella discussione della Commissione, possano davvero continuare a convivere ed a vivere attraverso il passaggio dell'Aula. Dico anche ai senatori che questo testo è molto in linea con la proposta di direttiva

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

un trattamento personale, connesso alla organizzazione e gestione delle prestazioni, gravemente degradante,

abbassare il limite ad un solo lavoratore occupato per quanto riguarda la chiusura dell'impianto.

non capisco la *ratio* che sta dietro al ragionamento, per altro, compiutamente argomentato. Allora, se la questione è questa, ossia che la clandestinità

la soluzione non può essere quella di incrementare le presenze irregolari, ma casomai, in un processo logico di ragionamento, esattamente l'opposto. Mi

questo non vuol dire - per essere chiari - trattare male le persone e non aver rispetto umano (questi sono altri ragionamenti), ma che, dal punto di vista del principio ideologico,

e non, come sempre, fare i forti con i deboli, quelli che le tasse le pagano già, girando la testa dall'altra parte, perché vi fa comodo, quando a commettere queste irregolarità sono quelli che volete difendere.

caso non c'era dubbio che sulla materia dello sfruttamento del lavoro servisse un intervento, e infatti mi pare che l'Unione Europea abbia forzato in questa direzione e abbia minacciato gli Stati membri addirittura di procedure di infrazione se non avessero ottemperato in tempi certi. Certo è che noi stiamo, come sempre, dimostrando di non sapere mai avere la bussola, di non sapere mai trovare la strada più equilibrata. Non c'è dubbio che per intervenire sulla codicistica penale, introducendo il grave sfruttamento e collegando il grave sfruttamento a sanzioni gravissime che comportano reclusioni da tre a otto anni, senza però capire che in ipotesi del genere potrebbero anche trovarsi persone che nulla hanno a che fare con lo sfruttamento del lavoro e dell'immigrazione,

bisognava provare ad anticipare, a prevenire. Stiamo parlando di reati legati allo sfruttamento dell'immigrazione e del lavoro nero, ma perché non pensiamo a come si crea il fenomeno dell'immigrazione e a come avviene il fenomeno della clandestinità nel nostro Paese? Questa maggioranza aveva un unico strumento che avrebbe consentito di controllare nel miglior modo gli accessi regolari nel Paese per non consegnarli alla malavita, come ha detto benissimo il mio collega.

combinava la permanenza sul territorio con un contratto di lavoro, cioè con la capacità di automantenersi. Il guaio è che adesso la si vuole cancellare, ma non solo: non è stata nemmeno applicata e si imputa alla mancata funzionalità ed efficacia della Bossi-Fini il fatto che questa debba essere soppressa. Vedremo prima se riuscirete a farla e poi quanti danni combinerà. tratta dell'unica legge che consentiva ad una persona d'arrivare in Italia e poter vivere dignitosamente con il proprio lavoro. Un

mosso da *pietas* cristiana, chiede ad un contadino se può provvisoriamente farsi carico di un disperato che si trova clandestinamente sul territorio italiano. Il contadino, stimolato dal prete di campagna, decide di farlo lavorare alle proprie dipendenze per fargli guadagnare un tozzo di pane. Ahimè, arriva il controllo e già con le norme che oggi esistono questo buon uomo con grande spirito caritatevole si ritrova in prigione. C'è di buono che il Paese fa quadrato, non c'è un biasimo sociale, ma c'è una certa solidarietà e ben o male questo signore, che è un imprenditore agricolo, riesce a uscirne indenne. Con questa norma, signori, non scapperebbe neanche più quello animato da *pietas* cristiana che si fa convincere da un religioso a fare un'opera caritatevole: rischierebbe addirittura da tre a otto anni di reclusione

vorrei comprendere da quali elementi i relatori e anche il Governo traggono la convinzione di sostanziale convergenza sulle disposizioni di questo disegno di legge. Sembra quasi che vi sia un'unanimità dell'Aula sulle disposizioni sottoposte alla nostra attenzione. Con altri colleghi, nel corso della discussione generale, abbiamo posto all'attenzione dei relatori e del Governo e anche della Presidenza alcune questioni che il Presidente della 1a Commissione ritiene serie - lo ha ribadito anche in questa sede -, prima fra tutte quella della sovrapposizione tra le disposizioni di questo disegno di legge e una parte della delega varata il 24 aprile dal Consiglio dei ministri, che attende ancora il passaggio nella Conferenza unificata Stato-Regioni. Io resto sorpreso nell'ascoltare anche in questa sede, come già è avvenuto nelle Commissioni riunite, l'argomentazione che ha adoperato il presidente Bianco, il quale ha detto che la questione era seria. L'abbiamo affrontata, abbiamo chiesto al Governo se, a fronte della sovrapposizione che è stata rilevata, intendeva andare avanti lo stesso con questo disegno di legge e il Governo ha detto che intendeva Noi abbiamo posto questioni di rilevo giuridico formale e sostanziale, riceviamo una risposta con un richiamo all'autorità, che nel caso specifico e in questo momento è - devo dire - l'assai problematico Governo in carica. Gradiremmo una risposta nel merito

che si sovrappone al contenuto di questo disegno di legge». Non mi accontento, signor Presidente, del fatto di dire che andiamo avanti. Che cosa significa andare avanti? Non è una risposta giuridicamente corretta e adeguata rispetto alle obiezioni che sono state sollevate. Nella discussione generale, ho l'impressione che i relatori abbiano tratto una valutazione di sostanziale convergenza da interventi da questa parte del Senato non totalmente ostili al disegno di legge. In realtà, abbiamo posto dei problemi. Vediamo in questo momento che i problemi sono accentuati

diventano disposizioni che illustrano un degrado e quindi rinviano ad un grave sfruttamento punito con pena da tre a otto anni di reclusione, con 9.000 euro di multa e con una serie di sanzioni accessorie che prevedono anche la chiusura dell'azienda. La nostra valutazione è fatta considerando i problemi posti sul tavolo che non hanno avuto risposte. Non abbiamo anticipato un giudizio sul voto finale, ma a questo punto il giudizio

facoltà. MANTOVANO *(AN)*. Spero che l'emendamento 1.101 non venga approvato e, signor Presidente, rivolgo un appello all'Aula in questa direzione. Tra le sanzioni accessorie rispetto a una norma, le cui ambiguità mi sono permesso di sottoporre all'attenzione dell'Aula prima, vi è anche quella in presenza dell'accertamento dell'occupazione di almeno tre lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale della sospensione delle attività dell'unità produttiva interessata per un mese. Dire a un'azienda che per un mese si bloccherà può essere una sanzione che svolge una funzione deterrente. Il parametro è di tre lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti. Questo emendamento addirittura propone

che possono essere accompagnate da intimidazioni che possono anche non essere tali e in più aggiunge, riducendo il numero di lavoratori necessari per l'applicazione di sanzioni accessorie, anche una simile pena accessoria. Se questo

anche legislativamente corretta comportamenti irregolari, con un giusto rapporto tra causa ed effetto, tra pena e colpa di chi si pone al di fuori della legge. Piuttosto, vuole sottolineare

sul discorso generale (che però è sempre collegato all'emendamento precedente), rilevando che questo incentivo all'immigrazione clandestina, che di fatto - ripeto - minimizza il reato di clandestinità,

Dirò di più. Innescate un circuito che invece di essere virtuoso è esattamente negativo al contrario. Con la vostra Con la vostra legge incentivate la presenza di persone irregolari che - ripeto - non arrivano su richiesta di una impresa o di una famiglia che hanno una necessità reale, ma anche un posto vero da occupare: semplicemente si immette sul mercato una quantità enorme di clandestini che poi, se vanno a lavorare clandestinamente, meglio, perché così diventano regolari. Voi incentivate la presenza di persone che a loro volta incentivano attività che di per sé sono o non regolari o comunque nella fascia più bassa della catena produttiva economica di valore aggiunto *pro capite*. Ripeto quello che ho detto prima: chi fa prodotti ad alto valore aggiunto, chi fa prodotti ad alta qualità, chi fa prodotti ad alta tecnologia, cioè esattamente le cose che con Bersani andate a dire in giro nei convegni, non ha bisogno del maghrebino irregolare che viene a schiacciare il bottone per tirare giù un pezzo di ottone da sbavare, ma impiega manodopera che evidentemente non può arrivare da tali situazioni. situazioni. In realtà, incentivate presenze massicce di persone irregolari a bassissima capacità professionale, che tengono in vita artificialmente la parte più bassa della nostra economia. economia. Fate l'esatto contrario di quello che andate a pontificare nei vostri incontri, nei vostri convegni o quando andate a parlare a Confindustria o agli imprenditori, perché la parte più bassa della tecnologia, quando non trova più manodopera, chiude e si rivolge alla parte più alta della tecnologia, dove trova la manodopera qualificata, con più esigenze ma che poi sa dare più valore aggiunto al prodotto finale. Queste sono le cose che voi - ripeto - pontificate, che andate ad osannare portando l'esempio della Finlandia che produce telefonini o degli altri Paesi nel mondo sviluppato che hanno trovato le nicchie ad alta tecnologia, ad alto valore aggiunto, ad alta qualità, e poi in Italia fate esattamente il contrario, ci riempite di persone che vengono qui già adulte e nei prossimi trent'anni o schiacceranno il bottone o sbaveranno le fusioni in fonderia o non sapranno cosa fare. Che logica c'è in questa cosa che andate a fare? Quella seguita nella legge Bossi-Fini di legare la necessità di queste persone all'effettiva disponibilità di lavoro nelle nostre aziende era l'unica modalità logica di gestire, dal punto di vista del lavoro, il fenomeno migratorio nel nostro Paese. Voi fate l'esatto contrario, condannando il nostro Paese non solo a restare per sempre nelle ultime posizioni di classifica tra i Paesi industriali, ma peggio, peggiorando artificialmente la nostra posizione, incrementando una situazione che di per sé non ci sarebbe. sarebbe. Se non ci fossero gli immigrati ma solo i cittadini italiani, infatti, l'industria si adeguerebbe alla manodopera disponibile in Italia, ma se riempite il Paese di milioni di persone senza professionalità fate l'esatto contrario. Se poi il problema che tirate fuori è che ci sono le famiglie lunghe grazie alla mentalità che continuate a perseguire contro la famiglia - che hanno bisogno di personale specifico nei servizi, come le badanti, è un altro discorso che non interessa milioni di persone che vengono per cercare lavoro, lavoro, ma eventualmente persone che arrivano da Paesi extracomunitari, come quelli dell'Europa dell'Est, molto più vicini a noi da un punto di vista culturale, e tutte le cose logiche e ovvie che potremmo dire, e che certo non disturbano il nostro Paese.

Con la scusa di fare quello che richiede l'industria italiana, mentre in realtà lo fate solo per questioni ideologiche ed elettorali, state facendo il male economico del Paese.

È utile che io parli perché se non utilizzassi il tempo che mi è consentito dal Regolamento in dieci minuti e quindi se non andassi oltre le ore 20 e l'emendamento fosse votato, il Governo potrebbe essere aiutato a non adire al detto latino *melius re perpensa*. Infatti, avendo votato l'articolo 1, quindi essendo stato esitato nella parte sostanziale il provvedimento,

questo provvedimento, non essendo un decreto e quindi non avendo effetti immediati per il Paese, non ha possibilità di essere approvato definitivamente, perché dovrà essere comunque varato dall'altro ramo del Parlamento. Quindi, si troverà in una sede istituzionale in cui contemporaneamente avranno

pensi il Governo, mediti sul fatto che i due emendamenti, quello precedentemente approvato e quello ora in esame, sono assolutamente vessatori e inaspriscono le

al Governo è - *melius re perpensa* - di non procedere al voto ed eventualmente di ritirare il provvedimento, perché ormai è chiaro, al di là della mia richiesta di non votare l'emendamento 1.101, che quest'ultimo non può essere votato.